Comunico che, in data 29 marzo 2016, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*: «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 14 aprile. L'ordine del giorno delle sedute di oggi è integrato con il prosieguo dell'esame del disegno di legge sul terzo settore. Rispetto agli altri argomenti già previsti dal precedente calendario dei lavori si aggiungono le ratifiche di accordi internazionali. Sulle relazioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti avrà luogo una discussione generale congiunta e seguiranno dichiarazioni di voto congiunte con attribuzione, a ciascun Gruppo, rispettivamente di dieci minuti per le fasi del dibattito. Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali risponderà a quesiti sull'attuazione e sugli effetti del *jobs act* e sulle prospettive di revisione della normativa pensionistica. Il calendario potrà essere integrato con informative del Governo sul caso Regeni e sui fatti di Bruxelles.

dallo Stato egiziano su questa vicenda, le chiedo di prevedere nel calendario non un semplice e generico riferimento alla possibilità che il Governo riferisca in Assemblea, bensì una data Propongo che mercoledì mattina della prossima settimana (quindi successivamente al giorno 5 aprile, quando, come abbiamo letto sulla stampa, ci sarà l'incontro degli investigatori),

le relazioni sul SIN di Porto Marghera e sul cosiddetto quadrilatero della chimica del Nord, si sta parlando non solamente di problematiche di natura ambientale (quindi, di conseguenza, anche di impatti negativi sulla salute umana),

Ci sono attività economiche che attendono da decenni la realizzazione delle bonifiche e della messa in sicurezza di questi siti, messa in sicurezza di questi siti, che non vengono realizzate per diverse responsabilità, ivi incluso il mancato finanziamento da parte del Governo.

è in grave difficoltà su questo tema. Siamo fortemente in ritardo sul *decommissioning* delle varie centrali nucleari che sono state spente dopo

con un costo eccessivo che aumenterà di anno in anno e che pagheranno tutti gli italiani sulla bolletta elettrica. Stiamo parlando di ritardi in ordine all'individuazione e alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi radioattivi e dell'assenza di un programma nazionale della gestione del combustibile nucleare, per il quale certamente arriverà a brevissimo l'ennesima e nuova procedura europea Stiamo parlando anche della mancata operatività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Il nostro Paese non è assolutamente protetto. Domani il *premier* Renzi si recherà a Washington per partecipare al *summit* mondiale sulla sicurezza nucleare e i tragici eventi degli ultimi giorni avvenuti a Bruxelles

del fatto che, per la vita e per la sicurezza del nostro Paese, è auspicabile che questa istituzione sappia farsi rispettare e pretenda che il Governo venga in Assemblea a render conto di ciò che sta facendo su questa materia. Non io, ma il Presidente del Consiglio europeo ha detto che l'accordo appena siglato tra Unione europea e Turchia avrà una gestione fallimentare

e che, nelle more dell'applicazione di quell'accordo, nasca una terza rotta: quella adriatica. Io credo che il Governo abbia il dovere di spiegare al Parlamento cosa intende fare e perché nell'accordo tra Unione europea e Turchia non ci sono elementi che diano garanzia a quella che, altrimenti, è la vittima designata di quest'accordo: mi riferisco all'Italia.

quali esiti stanno ottenendo, quali prospettive ha l'azione d'*intelligence* posta in essere, altrimenti non si capisce cosa ci sta a fare il Senato della Repubblica. La imploro, la prego, insisto perché si fissi una data certa in cui o il Presidente del Consiglio o il Ministro degli affari esteri o il Ministro dell'interno vengano in Aula e rendano conto alla Nazione (e non appena al Parlamento) degli errori, dell'approssimazione o quantomeno delle buone intenzioni (se ve ne da parte del Governo italiano di dare garanzie di sicurezza al nostro Paese. *(M5S)*. Signor Presidente, aggiungo qualche considerazione su questa richiesta. Il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede formalmente che il Governo

che vengano effettuate comunicazioni dell'Esecutivo sia sui fatti di Bruxelles, sia sul caso Regeni, sia sulla situazione della crisi mediorientale. Vogliamo che in quell'ambito i parlamentari, soprattutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle, possano presentare delle risoluzioni sulle comunicazioni del Governo, con parole scritte nero su bianco, in maniera da lasciare un atto di indirizzo al Governo e al ministro Gentiloni.

la discussione delle quattro relazioni della Commissione. Già c'era una contrazione nella discussione congiunta. Adesso i tempi contingentati renderanno difficilissimo affrontare i quattro argomenti differenti ed eterogenei che hanno interessato la Commissione finora e che sono stati portati a conclusione in queste quattro relazioni. Sfugge all'Assemblea l'importanza di questo dato, che è anomalo, in quanto non presente nelle precedenti legislazioni. È precisa volontà di questa Commissione

tutte e quattro le tematiche, dalla gestione dei rifiuti radioattivi alla questione delle bonifiche del polo chimico del quadrilatero del Nord (e nello specifico di Porto Marghera), ma finanche alla gestione dei rifiuti solidi urbani in territorio territorio ligure è che abbiamo una malagestione cronica, che serve a favorire gli illeciti. E questo Stato non vuole, non può o non ha ancora capito l'importanza di investire in sicurezza e gestione dei territori e del ciclo abbia presente le situazioni, anche perché il frutto del lavoro delle Commissioni d'inchiesta serve ai legislatori affinché si pongano rimedi alla normativa esistente attraverso la produzione Quindi, innanzitutto ritengo sia sfuggita all'Assemblea l'importanza e l'innovazione di questa proposta: me ne rammarico moltissimo e spero si possa tornare su questa decisione.

che, nella Conferenza dei Capigruppo della scorsa settimana, ha parlato di giganteschi investimenti nella sicurezza italiana. Ciò per noi è di vitale importanza, dato che i "giganteschi investimenti nella sicurezza italiana", nella scorsa legge di stabilità

Capisco che in questa Assemblea è difficile stare attenti alle esigenze dei cittadini, capisco che si può perdurare nel rallentare la soluzione delle esigenze dei cittadini italiani,

Vorremmo capire dal ministro Alfano che tipo e che livello di sicurezza verranno applicati nel nostro Paese, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi.

afferma che: «La fermezza e la dignità dei genitori di Giulio Regeni sono davvero esemplari. Motivo in più per le istituzioni per insistere con coerenza e altrettanta fermezza. Sulle risposte egiziane sentiremo in primo luogo le valutazioni del procuratore Pignatone».

il presidente dell'ultima Pro Loco dell'ultimo Paese d'Italia, ma il Ministro degli affari esteri, vorremmo capire - e questo Parlamento dovrebbe capire se affermazioni del genere sono stato fatte sull'onda dell'emozione di una giornata importante, come quella di ieri, o sulla base di un ragionamento politico ben preciso, da parte di un Ministro della Repubblica italiana.

*(LN-Aut)*. Insisto e, in caso di assenza di accordo, come si era già verificato, sulla votazione chiedo la verifica del numero legale.

all'articolo 6, vale a dire l'inclusione dell'impresa sociale tra gli enti del terzo settore. Ricordo che si tratta di enti che andranno a godere di agevolazioni consistenti - che non enuncio in questa sede, perché ne parleremo dettagliatamente all'articolo 9 e che dunque debbono avere finalità di tipo generale, sociale, con impatto su tutti i cittadini, e quindi, a nostro avviso, senza fini di lucro su tali attività. Qui abbiamo uno spartiacque tra chi crede che si possa fare mercato della solidarietà e del perseguimento della garanzia dei diritti sociali e civili e chi invece ritiene che ciò non sia possibile. Io sono dell'idea

con il «peloso» pretesto di perseguire anche una più piena occupazione. Ebbene, credo che proprio questo, invece, debba rimanere distinto, perché sui valori di solidarietà non si basa l'economia del Paese, ma si basano i principi di convivenza. le parole «e quindi» e di aggiungere questa imprescindibile precisazione: «L'impresa sociale non rientra negli enti del terzo settore». Diversamente dovremmo consegnarci progressivamente, oltretutto in una legge delega, alla volontà del Governo di favorire questa o quella impresa per interessi a volte anche meramente elettorali. Non sono concetti che esprimo solo io ma tanti enti, comitati, associazioni impegnate nel volontariato e che delle finalità solidaristiche sono pionieri da decenni.

di iniziativa governativa, purtroppo, ci sarà una maggioranza che vota compatta e una minoranza che difende dei principi.

territorio disseminato di iniziative virtuose; ma, nel momento in cui queste si aggregano, diventano facilmente parte della politica. Sappiamo che questo va evitato; quindi, limitare la dimensione economica di queste imprese non è solo un modo per limitarne la presenza sul mercato, ma è anche un modo per renderle più libere e più capaci di rispondere al reale benessere del territorio.

chiarire la finalità effettiva di questi enti. Laddove si prevede una remunerazione, è vero che facilmente entreranno dei soci privati, ma allora noi stravolgiamo il senso di queste imprese

sottolineare che deve essere prevalente la destinazione degli utili allo svolgimento dell'attività statutaria (che poi è stata peraltro modificata in "oggetto sociale"), è a nostro avviso un elemento di inquinamento. Lo diciamo con

prevedere in modo molto chiaro che non ci possono essere forme di remunerazione, se non quelle strettamente necessarie, come previsto per altri enti.

riferito alla destinazione degli eventuali utili alle finalità statutarie, non solo è sbagliato da un punto di vista concettuale, perché proprio le finalità di questi enti e la funzione

si realizzano, questi devono essere ricompresi totalmente nelle finalità dell'ente e non destinati ad altri usi, peraltro non diversamente specificati. Il testo arrivato in Il testo arrivato in Aula, quindi, non solo è sbagliato nel contenuto, ma è anche difettoso nel dare indicazioni su quali eventuali altre destinazioni possano possano essere ritenute accettabili. Questo testo è troppo vago e non può essere lasciato alla disponibilità del Governo, un domani.

Questo non può essere consentito in compresenza di remunerazioni del capitale, redistribuzione degli utili e perseguimento un fine di lucro. Va precisato almeno il rispetto del regime di libera concorrenza perché senza questo il dubbio che si stia cercando di fare dei favori indebiti non è più nemmeno un dubbio, ma una certezza.

Dal nostro punto di vista, la possibilità, nel rispetto delle disposizioni, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi d'amministrazione delle imprese sociali è irricevibile; va contro i principi di indipendenza dal potere politico che abbiamo poc'anzi espresso; va contro il principio che l'amministrazione del territorio debba vedere

cui si chiede semplicemente che gli enti pubblici e le organizzazioni private, che intendono accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale (cioè godendo di una forza lavoro gratuita), debbano possedere la caratteristica dell'assenza dello scopo di lucro. Se persone lavorano gratuitamente per svolgere un servizio sociale e civile,

una ipocrisia di fondo in questa norma o, meglio, nei potenziali decreti legislativi che ne discenderanno ma, soprattutto, ci esponiamo a incorrere anche in una violazione indebita del principio di concorrenza. Analogamente ciò accade per quanto riguarda la redistribuzione, ancorché parziale, con gli utili. Non è possibile ricevere qualcosa gratuitamente per ricavarne poi un vantaggio di tipo privato e privatistico.

è noto - il riferimento alle Province autonome estendibile all'interno del riferimento alle Regioni. Considero sostanzialmente recepito l'emendamento

Questo è il preludio agli altri emendamenti che abbiamo preparato, nel senso che l'attenzione da noi riservata all'articolo 8 va proprio nella direzione di far sì che le Regioni e le Province autonome abbiano una

potestà, da parte delle regioni e delle province autonome nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative» era proprio di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale, non compreso e non riconducibile all'articolo 52 della Costituzione.

si chiede che l'«allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui» diversi «territori regionali» sia equa e basata sui «principi di eguaglianza, pari opportunità, efficienza ed economicità» - potremmo considerarlo ovvio, ma nulla può darsi per scontato in una delega al Governo - e si utilizzino «criteri oggettivi, quali la percentuale di giovani residenti».

uno degli elementi che restituiscono ai nostri giovani la possibilità di accedere veramente a un diritto, oltre che a un dovere.

spontanea o istituzionale è fondamentale per la formazione dell'uomo e del cittadino. Ma quando si afferma che esperienze del genere debbano o possano essere valorizzate in ambito lavorativo, costituendo quindi titolo preferenziale nei concorsi pubblici - giacché questo non può valere nel campo privato, dove l'assunzione è discrezionale

Peraltro, il testo di legge non dice come verranno accreditati i soggetti che produrranno questi titoli da far valere come punteggio.

perché serve poi ad avere più facilmente accesso ad alcune professioni e, quindi, introduca il calcolo e la speculazione laddove dovrebbero esserci invece gratuità

la votazione perché "qui casca l'asino". Abbiamo cercato di escludere gli enti che perseguono fini di lucro e ridistribuiscono gli utili tra quelli che possono ricevere persone

che vi sia un concorso al finanziamento da parte degli enti che ne beneficiano. Se sono privati, hanno fine di lucro e possono ridistribuire gli utili, non è corretto che raccolgano gli utili

che non può essere quella di trasformazione in ordine del giorno, perché siamo già in legge delega. Ci deve essere un'assunzione di responsabilità per dire che almeno questo lo dobbiamo, veramente.

lo spirito della legge, vincolando il Governo a criteri, peraltro, minimamente restrittivi della facoltà di legiferare in maniera discrezionale, sono falliti. Sono falliti perché questa è la logica di quest'Assemblea, queste sono le logiche che regnano fuori da quest'Assemblea e che la svuotano spesso di significato. Il servizio civile universale era per me una grande occasione. Avrei voluto, anzi, estendere personalmente questa opzione, trasformarla addirittura in un qualcosa che fosse più vincolante e non solo premiato, ma addirittura proposto

fa scempio del patrimonio dei nostri padri, quelli che, uscendo dalla guerra, ancora avevano spazio, nel loro cuore e nella loro mente, per concepire qualcosa da fare a titolo gratuito per gli altri, dopo aver spezzato la schiena propria - e a volte quella dei familiari e dei figli - per portare a casa il pane per i propri cari. Ebbene, questo patrimonio qui viene sperperato, svilito. Avremmo voluto - ripeto - che questa fosse un'occasione. È un'occasione mancata e con sofferenza dovremo esprimere il nostro voto contrario. Presidente, voteremo contro l'articolo 8 perché già all'inizio era scritto in modo davvero bizzarro.

è finalizzato alla difesa non armata della Patria. Ora, mi chiedo come si faccia la difesa non armata della Patria, perché un conto è difendere i valori della Costituzione, altro è la difesa non armata: in che senso? Da che cosa? Mi sembra un tentativo di dare una vernice ideologica buonista, *politically correct*, finalizzata - questo sì - ad erogare un ennesimo finanziamento a qualche cooperativa, a qualche ONLUS ideologizzata, che magari già campa ampiamente di sussidi vari, in parte ricevuti, in parte estorti. A A questo si aggiunge l'accenno all'articolo 4, comma 2, della Costituzione, con riferimento al dovere di ogni cittadino di svolgere un'attività proficua per il progresso del Paese. Se, allora, è un dovere, deve essere accessibile a tutti. Come si fa a fare una cosa con bando al quale potranno accedere solo poche migliaia di giovani, facendo riferimento ad articoli della Costituzione che parlano del dovere? Se è dovere, è dovere dello Stato renderlo accessibile a tutti quanti, cosa che palesemente è impossibile. Si vuole allora fare tutta una bella salsa radical-progressista, *politically correct*, dove potranno guazzare le varie In questo senso erano giusti gli emendamenti che erano stati proposti perlomeno per escludere in modo esplicito le società - o qualsiasi ente che abbia scopo di lucro - dal poter avere

di questo servizio civile, per un verso perché avranno giovani che lavoreranno (in parte volontariamente, in parte con una sorta di rimborso spese a carico dello Stato) e Stato) e in più perché avranno una sorta di sanzione da parte dello Stato del loro ruolo straordinario. Peraltro, i giovani che andranno a prestare la propria opera gratuitamente

Qui stiamo davvero esagerando.

ho principi di fondo assolutamente antitetici a quelli del senatore Endrizzi, ma vedendo questo articolato arrivo alle sue stesse conclusioni. Io credo che qualsiasi impresa abbia un connotato sociale, dal laboratorio di una *start-up* di giovani studenti fino ad una multinazionale, perché un'impresa dà lavoro, produce beni e servizi per i cittadini e dunque ha un valore sociale. Proprio per questo ritengo che non ci dovrebbe essere una zona grigia tra le imprese di cui trattiamo in questa legge e quelle che rispondono ad una semplice logica di profitto. La differenziazione dovrebbe risiedere proprio nella certezza che le prime sono imprese volontarie, che rispondono alle stesse regole del capitalismo ma non per produrre lucro in termini personali. A me pare che questa legge non

e penalizzato quest'ambito, messa in evidenza dal senatore Marino, esce rafforzata e non indebolita dall'impostazione di questa legge. Per quanto riguarda poi il servizio nazionale svolto per la difesa della patria non in armi, questa è un'offesa per chiunque conosca un minimo la storia del secolo che è trascorso e non si faccia abbagliare da proposizioni che hanno un valore semplicemente ideologico. La difesa civile non in armi è stata compiuta dalle popolazioni che sono rimaste a casa, è stata fatta dalle donne, è stata fatta da quanti hanno resistito, sia nel corso della Prima, sia nel corso della Seconda, sia nel corso delle altre guerre, e non certo da qualche cooperativa

Signora Presidente, dichiaro il nostro voto a favore dell'articolo 8, perché per la prima volta, dopo tempo, si ritorna a parlare di servizio civile universale È una storia antica e travagliata, e vorrei ricordare tutta la vicenda legata all'obiezione di coscienza e quello che poi è seguito negli ultimi anni. Chi ha avuto l'opportunità, tra i giovani, di fare il servizio civile racconta di una grande opportunità umana solidale e culturale. Ritornare finalmente a parlare di servizio civile, dopo anni di oscurantismo, crediamo invece che sia molto importante. Certo, avremmo voluto un articolo molto più avanzato. Avremmo voluto - ad esempio - l'accoglimento del nostro emendamento sull'istituzione dei contingenti dei corpi civili un lavoro che ha la finalità di promuovere la prevenzione dei conflitti armati, la pace e la riconciliazione. Su questo punto abbiamo depositato uno specifico disegno di legge e proseguiremo con il nostro lavoro, perché per noi il dialogo interreligioso e la sicurezza umana intesa intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale, soprattutto nelle zone a rischio di conflitto armato, sono particolarmente importanti. Oggi dobbiamo dire che su questo continueremo il nostro lavoro e che

C'è un tema che riguarda ovviamente i finanziamenti, perché l'accesso al bando è legato ai finanziamenti che ogni anno il Governo stanzierà. Il Governo Renzi in merito aveva fatto degli annunci che poi non sono stati rispettati. Noi vigileremo, in maniera particolare in occasione della discussione

9.234 altrimenti il parere è contrario. Ho già detto alla collega Bignami che si tratta di una questione molto specifica

contrario

che svolgono un'attività commerciale non marginale. Dobbiamo pensare che la vendita di beni e servizi deve essere meramente occasionale, o comunque marginale dal punto di vista del valore economico, perché altrimenti non vedo come si possa rientrare nella definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, con tutte le agevolazioni che ne derivano, quando l'attività economica è consistente, se non addirittura prevalente. Noi dovremmo pensare che, così come definito nel testo attuale,

al Governo le direzioni lungo le quali procedere con i decreti legislativi.

una tassazione molto pesante e non è quindi pensabile che gli sgravi fiscali previsti all'articolo 9 (che magari elencherò in qualche prossimo intervento) vedano incluse

veramente abbondanti, almeno per gli impatti potenziali) presenti nell'articolo. Sappiamo benissimo che gran parte del finanziamento dei partiti avviene attraverso questi enti, che ufficialmente promuovono cultura ma che poi sostanzialmente promuovono questa o quella corrente politica, questo o quell'esponente politico. Se a questi enti diamo addirittura degli sgravi fiscali, noi stiamo finanziando in maniera surrettizia i partiti: questo deve essere chiaro. Non lo sto affermando io oggi, ma è stato detto in in tutti i modi dagli organi di stampa: anche organi di stampa di riferimento del PD come «la Repubblica» hanno denunciato quali e quante siano queste fondazioni e come esse rappresentino un sottobosco grigio che nasconde ai cittadini chi finanzia chi.

Presidente, mi riferisco a un fatto accaduto nell'ultima seduta dove, casualmente, era sempre lei a presiedere. Replicando a un mio intervento, il senatore Marton mi ha indicato come una persona che si permette di dire cose e e che, di fatto, non ha l'attendibilità per farlo, perché ha chiesto in lacrime di rimanere. A parte che non capisco dove io abbia chiesto di rimanere

il senatore Marton non era Capogruppo né ricopriva altro ruolo? Respingo pertanto l'accusa di inaffidabilità e dico che Marton è un bugiardo. Questa non è un'offesa, ma un dato di fatto perché, quando uno non riferisce riferisce le cose come stanno, è bugiardo e si qualifica per tale, come la maggior parte del Gruppo (non uniformo, però, perché ci sono dei notevoli distinguo da fare).

comportamenti assunti nei confronti di alcuni senatori, perché alcuni senatori sono stati impediti e inficiati nel loro mandato parlamentare. Signora Presidente, esattamente sette anni fa, il 30 marzo 2009, all'Aquila si riunì, per volere dell'allora capo della Protezione civile e sottosegretario Guido Bertolaso, la commissione grandi rischi. Quella commissione, dopo trentacinque minuti di riunione, per voce del vice capo della Protezione civile sentenziò che non c'erano pericoli incombenti, che la popolazione poteva stare tranquilla

del vice capo della Protezione civile, De Bernardinis, assolvendo tutti gli altri. Un vero e proprio capro espiatorio di una vicenda ben più complessa, che fu voluta dall'allora sottosegretario e capo della Protezione civile Guido Bertolaso, dal momento che lui stesso ammise, nelle intercettazioni telefoniche poi emerse, di voler fare esclusivamente un'operazione mediatica. Qualche giorno dopo quella riunione, il 6 aprile, una scossa terribile avrebbe ucciso 309 persone e distrutto migliaia di abitazioni. Parlo in quest'Aula per chiedere alla Presidenza del Senato di sollecitare la messa all'ordine del giorno della richiesta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'operato della commissione grandi rischi.

proprio per ricordare la beffa della finta riunione della commissione grandi rischi. Infatti, nelle motivazioni della sentenza relativa alla commissione grandi rischi,

la scorsa settimana, la compagnia aerea Alitalia-Etihad ha deciso di sopprimere il collegamento tra Roma e Pescara, introdotto poco più di un anno fa,

ci sarà inevitabilmente un peggioramento del trasporto pubblico e un maggiore isolamento dell'Abruzzo, soprattutto sull'asse Est-Ovest del Paese, con gravi ripercussioni sul turismo e sul tessuto economico di una Regione che, ormai da troppi anni, registra una perdurante crisi economica,

aeroportuale italiano, con particolare riferimento proprio all'aeroporto di Pescara, che solo nel febbraio 2015 era stato considerato come scalo di interesse nazionale. Inoltre, chiedo al Ministro di promuovere un tavolo di concertazione con la Regione,

Le richieste in questione sollevano una situazione di anomalia nei trattamenti nei confronti di molti lavoratori, che assomiglia molto al *mobbing* di gruppo e che ancora ancora oggi si sta verificando al cantiere nautico Nuovi cantieri Apuania (NCA) di Marina di Carrara. A partire dal gennaio del 2015, 43 lavoratori hanno subito un sistematico processo di emarginazione, condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali, indispensabili allo svolgimento della normale attività Dopo le prime due interrogazioni, alle quali questo Governo non ha risposto, abbiamo fatto richiesta di documenti al Ministero dello sviluppo economico (MISE) per visionare gli atti completi di acquisto da parte dell'acquirente di NCA, cioè la società Moda design, dell'imprenditore Giovanni Costantino. Non avendo avuto risposta, abbiamo ulteriormente inoltrato

per avere un briciolo di attenzione da parte di questo Governo. Ora il problema è che ancora ad oggi nella società NCA persistono le vessazioni nei confronti di questi lavoratori. Non solo, la proprietà non si accontenta più di umiliarli, ma è passata alla fase 2, chiedendo la mobilità per 40 lavoratori contrariamente agli accordi stipulati al Ministero, per i quali si impegnava a riassorbire 105 lavoratori in cambio di agevolazioni incredibili, compresa la cessione trentennale del suolo demaniale. Per ottenere ciò, l'imprenditore Giovanni Costantino doveva ricollocare in due fasi i 105 lavoratori di NCA nella nuova impresa, ma pare che rispettare i patti sottoscritti per qualcuno sia un *optional* o una "gentile concessione". Gli esuberi dei 40 lavoratori che oggi l'azienda annuncia non stanno né in cielo né in terra. Il piano industriale non è mai stato presentato chiaramente e ciò che è stato stipulato, per esempio le nove commesse annuali, sono promesse di Pulcinella. Lo smantellamento

A chi giova tanta magnanimità? Ai lavoratori certo no!Alla certezza del lavoro certo no! Allo sviluppo del territorio certo no! Quindi da quest'Aula invito tutti coloro che anche nella mia zona si stanno stracciando le vesti per tutelare il diritto del lavoro, magari politici e che magari sono in partiti di maggioranza, a sollecitare il loro Governo renziano affinché risponda alle nostre innumerevoli interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni. Abbiamo bisogno di risposte vere e concrete. L'aria la porta via il vento, gli atti restano. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza per rassicurare tutti questi lavoratori del cantiere NCA. Il Governo risponda. Non è più tempo di tacere o di scansarsi dalle responsabilità. **Mozioni,